gli ottimi abitanti di Fondi purtroppo hanno una complicata amministrazione comunale, che è stata oggetto di ripetute richieste di scioglimento da parte del Ministro dell'interno; ancora in un *question time* recentissimo, il Ministro dell'interno ha sollecitato lo scioglimento del Consiglio comunale.

di impiegati nei Consigli comunali i giocatori di calcio. Mi sembra che questa vicenda sia di particolare gravità; comunque, c'è un reato evidente. Non so cosa mi risponderà il Governo, ma una cosa è certa:

ma soprattutto credo che si debba passare ad una vera e propria trasmissione di atti per un'incriminazione quantomeno per peculato per distrazione.

che le disposizioni federali, in ossequio a quanto previsto dalla legislazione statale, consentono di riconoscere ad atleti dilettanti soltanto i rimborsi spese, le indennità di trasferta ed eventuali premi partita. Pertanto, ulteriori accordi economici in contrasto con le suddette norme non sono consentiti ed espongono le società ed i tesserati a sanzioni disciplinari. Con specifico riguardo alla predetta società "Football Club Fondi", si fa presente che la Federcalcio, acquisita ogni opportuna informazione sui tesseramenti della società direttamente dal comitato regionale Lazio della Lega nazionale dilettanti, ha comunicato che il parco calciatori attualmente in carico alla società Fondi è formato da 55 tesserati, di cui cinque hanno militato in categorie professionistiche negli anni scorsi, e non risultano calciatori ex professionisti tesserati con la società Fondi per la prima volta nella stagione sportiva 2008-2009. La Federcalcio ha anche precisato che è consuetudine che alcuni ex professionisti, nella fase finale della carriera, continuino a giocare in categorie inferiori e quindi anche in quelle dilettantistiche. Con riguardo alla richiesta degli onorevoli senatori interroganti, si fa presente che l'acquisizione di informazioni sul comportamento degli enti ed organismi pubblici, affidata ai Servizi ispettivi di finanza pubblica, ha la finalità di verificare l'andamento delle spese e dei bilanci di tali organismi allo scopo di assicurare il perseguimento degli obiettivi di finanza pubblica. Tali accertamenti sono strumenti di controllo privi di poteri coercitivi e sanzionatori, che esauriscono di norma i loro effetti entro la sfera delle attività referenti, demandando alla competenza degli enti e delle amministrazioni interessate l'adozione dei provvedimenti correttivi sulla sulla base dell'esito degli accertamenti eseguiti. Si precisa, infine, che il Ministero dell'economia e delle finanze, considerato il numero di segnalazioni che pervengono su questioni riguardanti gli enti locali, in sede di programmazione annuale seleziona le segnalazioni che presentano particolari criticità ed al fine di un eventuale inserimento nel programma ispettivo valuta se le problematiche segnalate sono compatibili con gli obiettivi fissati dalla direttiva ministeriale sull'azione amministrativa cui la programmazione annuale si ispira. È in quest'ambito, pertanto, che sarà valutata la situazione riferita con la presente interpellanza.

essa riguarda soltanto la sfera della regolamentazione del rapporto sportivo. In questo caso, c'è una *mala gestio* amministrativa: il Consiglio comunale prende i soldi dei cittadini di Fondi e ci paga i calciatori. Ma siamo matti? Mi riservo, con la copia della risposta, di intervenire ancora presso altro Ministero.

A seguito di quanto disposto dalla legge 14 agosto 1991, n. 281 (Legge quadro in materia di animali di affezione e prevenzione del randagismo), tutte le Regioni e le Province autonome hanno attivato la rispettiva anagrafe canina e ne hanno reso possibile la consultazione per via telematica. Al fine di ribadire la necessità dell'identificazione e della contestuale registrazione dei cani, è stata emanata l'ordinanza ministeriale 6 agosto 2008, che dispone, tra l'altro, l'interoperatività delle anagrafi canine regionali con quella nazionale, alla quale devono essere trasmessi i necessari flussi di aggiornamento. Per quanto riguarda il risanamento dei canili e la costruzione di nuovi rifugi per i cani, la stessa legge prevede un fondo annuale per la lotta al randagismo, utilizzato anche per la realizzazione delle citate opere; inoltre, la legge 29 dicembre 2003, n. 376, concernente «Finanziamento di interventi di opere pubbliche», ha previsto un finanziamento *ad hoc*. Sono peraltro consapevole che la costruzione dei canili e dei rifugi non è sufficiente per una lotta fattiva al randagismo, come io la intendo, se non è accompagnata, tra l'altro, da un'assunzione reale di responsabilità amministrativa da parte delle Regioni e dei Comuni e da un'adeguata preparazione di tutte le figure coinvolte nella tutela degli animali. A tal proposito, questo Ministero sta ultimando, proprio in questi giorni, la predisposizione di un disegno di legge del Governo per la tutela degli animali d'affezione e per la prevenzione e il controllo del randagismo. Il disegno di legge, che è innovativo, prevede, tra l'altro, la formazione dei gestori dei canili, dei proprietari e degli allevatori; riunisce le ordinanze emanate e che hanno quindi scadenza; sviluppa, in un quadro più articolato e complesso, quanto già parzialmente anticipato con la recente "ordinanza contingibile ed urgente concernente la tutela dell'incolumità pubblica dall'aggressione dei cani". Inoltre, con il suddetto disegno di legge verranno recepiti nel nostro ordinamento giuridico anche quegli aspetti della Convenzione di Strasburgo del 1987, che purtroppo sono rimasti finora disattesi. Relativamente alla ratifica della Convenzione del Consiglio d'Europa di Strasburgo, il 29 gennaio 2009 si è tenuta una riunione di coordinamento presso il Ministero degli affari esteri circa le modalità e i tempi necessari. Segnalo che questa Amministrazione ha ultimato la predisposizione del disegno di legge per la ratifica (che prevede anche il divieto di mutilazioni e le sanzioni per il reato di importazione clandestina dei cuccioli), di cui si auspica un sollecito *iter* parlamentare. Per quanto riguarda le iniziative adottate, preciso che, per contrastare l'inerzia di alcune amministrazioni locali, questo Ministero ha disposto una serie di ispezioni nelle Regioni che presentano le situazioni più critiche. Inoltre, nell'ambito della campagna ministeriale per la tutela degli animali d'affezione, avviata nel mese di luglio 2008, il Comando dei Carabinieri per la tutela della salute (NAS) ha effettuato, su tutto il territorio nazionale, ispezioni circa le attività di allevamento, addestramento, ricovero e vendita di cani e le corrispondenti strutture. Inoltre, in merito alla grave situazione esistente nella Regione Sicilia, culminata con i fatti di Scicli e Modica, preciso che l'intervento degli ispettori veterinari della direzione generale competente è stato immediato e supportato da un intenso lavoro di collaborazione, peraltro ancora in atto, con le autorità sanitarie regionali. È stato predisposto un "Piano straordinario randagismo" che, già avviato nella Provincia di Ragusa, sarà poi attuato con i relativi aggiustamenti in tutta la Regione, costituendo, inoltre, un modello esportabile su tutto il territorio nazionale.

Ribadisco la necessità che tutte le istituzioni locali si adoperino concretamente nella lotta contro il randagismo, sia per l'incolumità pubblica sia per evitare il ripetersi di episodi di violenza ingiustificata contro i cani randagi, sia per prevenire patologie trasmissibili dall'animale all'uomo. Il Piano, che prevede la collaborazione delle associazioni animaliste, consiste in una serie di iniziative che ricomprendono l'anagrafe canina, con l'identificazione e la registrazione massiva dei cani di proprietà, e le sterilizzazioni che saranno a carico del Servizio sanitario nazionale; i cani verranno poi collocati in strutture rifugio il cui numero dovrà essere potenziato. Sarà anche prevista l'incentivazione delle sterilizzazioni dei cani di proprietà, in particolar modo di quelli presenti nelle aree rurali o suburbane. Nel Piano viene sottolineata l'importanza anche di una campagna di informazione e dei corsi di formazione, da avviare nelle scuole, per sensibilizzare i giovani e in generale i cittadini al rispetto verso questi animali. In merito alla verifica dell'impiego dei fondi stanziati per prevenire il fenomeno del randagismo, va precisato che il decreto interministeriale del 6 maggio 2008, recante "Criteri per la ripartizione del fondo per l'attuazione della legge n. 281 del 1991", obbliga le Regioni e le Province autonome a inviare al Ministero una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente. Intendo sottolineare che le iniziative adottate finora dal Ministero rappresentano solo la preliminare fase d'avvio per garantire la completa applicazione sul territorio nazionale della normativa vigente in materia di salute e benessere animale,

Gentile Sottosegretaria, le sua informativa è interessante e sicuramente apprezzabile. Questo evidentemente non ci consente di dichiararci soddisfatti, come credo non sia soddisfatta lei, conoscendo la sua disponibilità e la sua attenzione personale ai temi che riguardano gli animali da affezione. Credo che alcuni passi si stiano compiendo, ma con una lentezza istituzionale a mio avviso inadeguata alla situazione purtroppo naturalmente abbastanza complicata e grave già esistente in Italia. Siamo convinti che il lavoro avviato sia positivo; tra l'altro, c'era una disponibilità dichiarata, non solo a parole, da parte delle forze di opposizione, e non solo, a lavorare insieme per arrivare presto nelle Aule parlamentari a modificare quelle leggi che, pur ottime, si sono dimostrate ormai vetuste, quindi necessitanti di essere aggiornate. Mi riferisco alla legge contro il randagismo e a quanto ad essa è

la nostra reciproca attenzione i casi di violenza sugli animali perpetrati anche da bambini, come la vicenda del ragazzino di nove anni che non solo ha seviziato e ucciso un piccolo animale, ma ha anche fatto riprendere l'episodio e l'ha messo in rete; quindi, temi che riguardano l'educazione, peraltro già previsti dalla legge n. 189 del 2004, e non solo. Si tratta di capire come riusciamo poi, nella pratica, a dare attuazione a questi elementi assolutamente non secondari. Ad esempio, noi pensavamo che per quanto riguarda il controllo, in particolare delle Regioni, l'inserimento nell'elenco degli obiettivi di valutazione dei direttori delle aziende sanitarie locali anche degli aspetti che riguardano la prevenzione del randagismo e il benessere animale potesse essere un elemento utile, perché sappiamo che spesso di queste cose poi ci si occupa solo in apparenza e non nella sostanza, altrimenti alcuni elementi

perché ormai sono trascorsi più di vent'anni e recepirla sarebbe un dovere. Quindi, comprensione, anzi condivisione, per quelle questioni che insieme, dal punto di vista culturale ed umano, sappiamo essere sentite.

Sappiamo che non ci sono bacchette magiche. Riconfermiamo pertanto la nostra piena disponibilità per arrivare, però in tempi veloci, ad atti legislativi concreti, che finalmente consentano al nostro Parlamento non solo di dichiarare, ma anche di varare

avere per tre anni quasi 5 milioni di euro in meno rispetto a quanto le Regioni, i Comuni e le società di volontariato ritenevano di poter disporre è un qualcosa che mette noi tutti in un'affannosa salita. chiedere cosa fare in una simile situazione. Le iniziative legislative che il Governo ha proposto ci vedono - come ha detto la senatrice Amati - partecipi, attenti. Contribuiremo, valuteremo e non avremo nessuna difficoltà a dire: bene, molto bene.

e anche, nell'attesa di una nuova cornice legislativa, potenziando la prassi del confronto e delle migliori pratiche e una cooperazione tra le città più virtuose e le realtà che hanno maggiori difficoltà.

di confronto per verificare se il coordinamento legislativo non è puramente formale ma è tale da incidere su una realtà che sta diventando davvero molto fragile e pericolosa, specialmente a fronte di risorse decrescenti nei prossimi anni.

che, nell'immediato, il competente compartimento ANAS di Bologna, d'intesa con la Protezione civile, con la Provincia e il Comune, ha individuato un percorso alternativo provvisorio in corrispondenza del vecchio tracciato della statale, non utilizzato dagli anni Settanta, al fine di consentire il collegamento con i minimi requisiti di sicurezza. Conseguentemente, sono state avviate tutte le attività necessarie a ripristinare rapidamente il collegamento delle frazioni Cerreto Alpi e Cerreto Laghi con il resto della provincia reggiana. Si è in tal modo provveduto, mettendo in atto interventi di disboscamento e pulizia delle opere idrauliche, rimozione del materiale detritico lungo il vecchio tracciato della statale 63 dal chilometro 44,100 al chilometro 42,900 e il movimento di terra necessario al ripristino della viabilità; è stata altresì disposta la fornitura e posa in opera di rete metallica per il rivestimento di pareti e scarpate, pannelli, funi e chiodature e, infine, di consolidamento della frana in corrispondenza del raccordo di monte del vecchio tracciato con la strada statale 63 mediante gabbioni, ripristino pavimentazione del vecchio tracciato e posa in opera di barriere di sicurezza. Nonostante le avverse condizioni meteorologiche e le notevoli problematiche che presentava il vecchio tracciato, l'ANAS ha ripristinato il collegamento in meno di due settimane, evitando disagi ai residenti in previsione delle festività natalizie. Contestualmente, è stato istituito un tavolo tecnico di coordinamento tra ANAS e Protezione civile dell'Emilia-Romagna. Il monitoraggio, disposto e seguito dalla Protezione civile e dalla Difesa del suolo della Regione, che sono i soggetti istituzionalmente responsabili per il controllo della stabilità dei versanti, è attualmente in corso e consentirà di acquisire i dati per controllare il percorso alternativo appena ripristinato e quelli utili ad individuare gli interventi definitivi da adottare per il ripristino della viabilità principale della statale 63. I risultati delle indagini che scaturiranno da tale monitoraggio consentiranno, pertanto, di stabilire i tempi e gli importi necessari all'esecuzione dei relativi interventi. Il progetto atto a migliorare le condizioni di sicurezza del percorso provvisorio attuale è stato redatto ed approvato in linea tecnica. Lo scorso 12 giugno è stato pubblicato il bando di gara per l'affidamento dei lavori di pavimentazione e di protezione del corpo stradale sul tratto della statale «del valico del Cerreto» interessato dai movimenti franosi. L'importo dei lavori, finanziati da ANAS, è di 1,5 milioni di euro.

che il cedimento viario di cui stiamo discutendo interessa il cuore di questo territorio e lo ha in qualche modo spezzato in due. Per giorni - come lei ricordava, signor Sottosegretario - l'interruzione ha isolato le frazioni di Cerreto Alpi e la stazione sciistica di Cerreto Laghi

Abbiamo visto la Regione assumersi l'onere di finanziare e realizzare assieme alla Provincia l'indagine geognostica e i monitoraggi necessari a comprendere la portata del fenomeno: trattasi di 210.000 euro, con indagini che si stanno avviando.

studia anche possibili alternative e, assieme alla Provincia di Massa, sottoscrive un accordo per l'ipotesi di un tunnel che colleghi maggiormente i due versanti. Vista l'importanza di tale asse e il rischio di tenuta dei territori montani interessati, che sulle comunicazioni giocano gran parte del loro futuro, credo che il Governo non si sia attivato adeguatamente ed abbia affrontato genericamente l'emergenza.

la linea ferroviaria Brescia-Parma è stata interrotta al traffico ferroviario nella tratta tra le stazioni di Torrile San Polo e di Parma a partire dal 14 giugno 2004, per consentire i lavori finalizzati alla costruzione dell'interconnessione di Parma tra la nuova linea ferroviaria ad alta velocità-alta capacità Milano-Bologna e la linea storica. La linea, con esercizio a trazione diesel, è lunga complessivamente 92 chilometri da Brescia a Parma, di cui 7 chilometri di tracciato, dalla stazione di Brescia a quella di San Zeno-Folzano, sono comuni alla linea Brescia-Cremona. Le stazioni e le fermate intermedie tra Brescia e Parma sono 16, mentre nella stazione di Piadena la linea si affianca a quella Codogno-Cremona-Mantova. Non esistono stazioni o fermate intermedie tra quelle di Parma e di Torrile San Polo, che distano 10 chilometri l'una dall'altra, e sono oggi i capolinea del tratto ferroviario interrotto dove si attesta il servizio di bus sostitutivo gestito da Trenitalia. A seguito dell'interruzione succitata, i collegamenti nella tratta Torrile San Polo-Parma sono stati riorganizzati attraverso servizi sostitutivi con autobus. Sulla relazione Torrile San Polo-Parma (e viceversa) sono attualmente previsti, in un giorno feriale medio, 26 servizi effettuati con bus (che trasportano circa 11.000 viaggiatori a settimana), con tempi di percorrenza su strada che vanno dai 20 ai 30 minuti (a seconda della fascia oraria e, quindi, dell'intensità del traffico stradale). Gli autoservizi effettuano le medesime fermate dei treni che sostituiscono e i relativi orari sono programmati in modo da assicurare le coincidenze con il servizio ferroviario. La pianificazione e l'avanzamento delle attività di realizzazione dell'interconnessione di Parma Est e di modifica del PRG della stazione di Parma, sia per quanto riguarda le attività di competenza del *General Contractor*, sia per quelle di competenza delle Direzioni compartimentali infrastruttura di Rete ferroviaria italiana di Milano e di Bologna, hanno consentito di pianificare la riattivazione delle tratta interrotta Parma-Torrile San Polo, e della linea Parma-Suzzara,

la risposta all'interrogazione, che mi lascia ovviamente parzialmente soddisfatto, perché viene comunque indicata la data del

vengano tenute presenti sia nell'azione del Governo che nelle proposte e nell'attenzione del Parlamento.

tra i vari progetti di Rete ferroviaria italiana in Sicilia, attualmente a diversi stadi di avanzamento destinati ad aumentare e migliorare la capacità e la funzionalità della rete nella Regione, è da segnalare sulla linea Palermo-Messina il raddoppio della tratta Fiumetorto- Ogliastrillo-Castelbuono. Il raddoppio di circa 32 chilometri è previsto parte in affiancamento da Fiumetorto a Lascari, e parte in variante in galleria da Lascari a Castelbuono

Nel 2005 sono state consegnate le prestazioni al *General* *Contractor* per la realizzazione degli interventi nella tratta Fiumetorto-Cefalù Ogliastrillo. Dopo lo sviluppo della progettazione esecutiva da parte del l'apertura dei cantieri è avvenuta il 13 maggio 2008. L'attivazione della tratta Fiumetorto-Ogliastrillo è invece programmata nel 2011. Il contratto di programma 2007-2011 (aggiornamento 2008), siglato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dalla Rete ferroviaria italiana, include il progetto del «Raddoppio Palermo-Messina» in tabella A04, «Opere in corso», con un costo complessivo di 1.672 milioni di euro circa, di cui: 728 milioni per il raddoppio della tratta Patti-Messina, compreso il Sistema di comando e controllo della circolazione; per la realizzazione della tratta Fiumetorto-Ogliastrillo; 530 milioni per la realizzazione della tratta Ogliastrillo-Castelbuono, compresa la realizzazione della nuova fermata in galleria di Cefalù. Questa tratta, per carenze di finanziamenti in termini di cassa, nel citato contratto è previsto da realizzare oltre l'arco di Piano. Per dare impulso a tale tratto di raddoppio, nell'ambito dell'aggiornamento 2009 del contratto di programma 2007-2011 si sta verificando la possibilità di anticipare la realizzazione dell'opera; su tale base si può ipotizzare l'affidamento dell'appalto principale nel primo semestre del 2010.

Sulle infrastrutture si fa un gran parlare: promesse, annunci, convegni ed anche aperture di cantiere che spesso non corrispondono alla realtà. Addirittura, a fine 2008, per dare una risposta alla crisi si è parlato di un investimento da parte dell'attuale Governo sulle infrastrutture nel Mezzogiorno d'Italia di 16 miliardi di euro. I fatti invece non ci dicono questo. Ci parlano invece di un'assenza di interventi reali e concreti. Prendiamo l'esempio della linea ferroviaria Palermo-Messina.

si tenterà di anticipare al primo semestre 2010. Caro Sottosegretario, così non si può procedere. E' importante invece cambiare passo, essere seri e fare in modo che quando si guarda un'opera pubblica innanzitutto si interviene per cassa; luogo, si interviene immediatamente. Tutti sanno che queste due tratte debbono procedere insieme perché se va avanti una e non si fa l'altra, caro Sottosegretario, si creeranno solo delle disfunzioni.

che hanno dimostrato che queste opere si possono fare, si possono fare bene e vanno insieme; 32 chilometri da fare insieme. Avevate una grande opportunità. Invece, in questi mesi, avete tolto risorse alle infrastrutture in Sicilia.

dei soldi che non sono stati utilizzati da Agenda 2000-2007; oppure, potreste intervenire su Agenda 2007-2013. Anche qui, nessun segnale! Anzi. Voi sapete che c'è un contenzioso rovinoso,

per cui sono negate delle risorse fondamentali che potrebbero essere utilizzate per veri investimenti, cantierabili ed in grado di dare risultati importantissimi. Ecco perché non sono per niente soddisfatto. Ecco perché, accanto a questa mia insoddisfazione, ho avanzato delle proposte. La prima: smettetela di fare ancora degli annunci. Mettetevi sul serio al lavoro. Evitate che le vostre lotte intestine producano danni alle infrastrutture in Sicilia. Utilizzate le risorse che avete annunciato; poi, siccome non le avete realmente, almeno utilizzate quelle di Agenda 2000-2007 o quelle di Agenda 2007-2013. Fate in modo che la programmazione non sia sconnessa, con i lavori già partiti per la prima tratta. La prima tratta darà delle risposte, la seconda no. Ecco perché è importante che cambiate passo. Questo Governo la smetta di fare annunci sulle infrastrutture: cominci a lavorare sul serio, a cooperare con le realtà territoriali, con le Regioni.

in data 21 maggio ultimo scorso, nelle prime ore del mattino, si è verificato, lungo la strada statale 626 Caltanissetta-Gela, un cedimento del piano viabile in corrispondenza del giunto posto sulla pila n. 11 del viadotto "Geremia 2". Il viadotto è stato immediatamente interdetto al traffico in entrambe le direzioni e la circolazione è stata deviata sulla strada provinciale n. 18. L'ANAS ha quindi nominato una commissione tecnica interna, coadiuvata da docenti universitari, con il compito di stabilire le cause dell'evento, la congruenza delle opere realizzate con il progetto e la soluzione per il ripristino definitivo della struttura. Contemporaneamente, la procura di Gela ha avviato un'indagine sull'accadimento, disponendo il sequestro dell'area ed apposita CTU per individuare le cause. Nelle more dell'autorizzazione, richiesta da ANAS alla magistratura per effettuare opere di pronto intervento per una prima messa in sicurezza del viadotto, si è verificato un ulteriore movimento della predetta pila, con il conseguente crollo dell'impalcato appoggiato sul lato Gela. La commissione tecnica ANAS ha proceduto e sta procedendo, oltre che ai necessari accertamenti - l'ultimo è stato effettuato l'11 giugno - a predisporre un programma di sondaggi, carotaggi e rilievi finalizzati ad individuare le cause dei citati fenomeni

rispetto alla quale questa società ha nominato due tecnici interni ed un docente di geotecnica dell'università di Napoli, quale consulenza tecnica di parte.

Sottosegretario, al di là delle spiegazioni che sono state fornite oggi in Aula, rimane assolutamente incomprensibile proprio quanto è accaduto, è accaduto, in due distinti momenti e nell'arco di una settimana. Infatti, così come lei ha detto, nel maggio del 2009, lungo la strada statale 626 Gela-Caltanisetta, niente è andato per il verso giusto secondo le regole e le procedure di quello che viene definito un Paese moderno.

un quadro fosco, che, senza anticipare ‑ non credo sia possibile ‑ le conclusioni della magistratura permette di preconizzare una grave responsabilità da parte di chi ha costruito il viadotto "Geremia 2" e di chi non ha effettuato i necessari controlli. La piaga del calcestruzzo debole o difettoso si sta mostrando in tutta la sua ampiezza nell'ambito regionale siciliano. Mi auguro perciò che siano presi opportuni provvedimenti. L'interrogazione presentata richiedeva che lei entrasse

certamente non una consolazione adoperarli in questa direzione. Si parla, infatti, di risorse che in nome di una perenne logica emergenziale verranno certamente sottratti allo sviluppo della Sicilia. Ecco perché non posso assolutamente dichiararmi soddisfatto, non solo delle risposte che sono state date, ma soprattutto di ciò che immagino dovrà avvenire tra poco quando ancora una volta recupereremo quei dati da cui emergerà come siamo stati sbeffeggiati da controlli che non sono stati sapientemente fatti.

telecomunicazioni. Nasce dalla fusione di Alcatel e Lucent Technologies. Occupa in Italia circa 2.300 lavoratori nelle proprie sedi situate a Vimercate, Trieste, Genova, Roma, Rieti, Bari e Battipaglia. A seguito della notizia di un progetto di chiusura dello stabilimento di Salerno da parte dell'Alcatel, su sollecitazione delle parti coinvolte dalla vicenda, mercoledì 29 maggio 2009 si è tenuta presso il Ministero dello sviluppo economico una riunione riguardante lo stabilimento di Battipaglia dell'Alcatel-Lucent. Alla riunione hanno partecipato oltre ai rappresentanti del Ministero che rappresento, rappresentanti del Ministero degli esteri, del Ministero del lavoro, della Regione Campania, e dell'azienda, unitamente alle organizzazioni sindacali di categoria nazionali e territoriali e alle RSU aziendali. alle RSU aziendali. Lo scopo di tale incontro è stato avere conferma delle reali intenzioni della multinazionale francese sul citato stabilimento. Nel confronto tenutosi presso il Ministero dello sviluppo economico, il rappresentante dell'azienda ha sottolineato che, a fronte della sollecitazione del Governo e delle organizzazioni sindacali, è stata chiesta alla direzione di Parigi una lettera che chiarisse le posizioni del Gruppo in Italia. Il direttore delle attività dell'Alcatel-Lucent dell'Alcatel-Lucent per l'Europa, il Medio Oriente e l'Africa ha indirizzato una missiva alle organizzazioni sindacali italiane in cui conferma il ruolo strategico per l'Alcatel delle proprie attività in Italia. La cessione della parte produttiva di Battipaglia va inserita, pertanto, nell'ambito della strategia globale del Gruppo che punta ad ottimizzare la propria organizzazione. Ciò non influirà, tuttavia, sulle attività del sito, riconosciuto dalla proprietà come centro di eccellenza globale. La politica di razionalizzazione delle attività dell'intero gruppo Alcatel-Lucent prevede la riduzione dei lavoratori interinali, soluzione che avrebbe consentito al sito italiano di restare attivo, anche se con un organico ridotto. Si sarebbe trattato comunque di una soluzione temporanea: per ogni area geografica, il gruppo prevede infatti la presenza di un solo centro produttivo; in Europa, sarà ovviamente quello francese. Ha aggiunto infine che mantenere l'attività ed il sito di Vimercate rappresenta quindi già un'eccezione rispetto a quanto previsto dai vertici dell'azienda. Sul sito di Battipaglia sono stati prospettati due scenari. Il primo prevede la riduzione del numero dei lavoratori interinali e porterebbe il totale degli occupati a circa 80, parte dei quali continuerebbe a lavorare con la R&D, mentre un'altra si dedicherebbe alla produzione; ulteriori 30 persone potrebbero inoltre accedere al trattamento pensionistico e ciò ridurrebbe sensibilmente il numero degli occupati mettendo a serio rischio la continuità del sito. Il secondo scenario invece prevede, con la collaborazione delle parti interessate, l'elaborazione di un progetto che consenta di mantenere la produzione per un periodo prefissato a Battipaglia, per dare continuità operativa al sito e salvaguardare anche i lavoratori interinali. L'azienda ha dato la propria disponibilità a discutere entrambe le possibilità. Le organizzazioni sindacali hanno fatto notare come la produzione di Battipaglia possa rivelarsi strategica nei prossimi anni, anche in relazione ai progetti pubblici relativi alla banda larga e hanno inoltre fatto presente che le organizzazioni sindacali aziendali hanno proposto un progetto che potrebbe consentire la sopravvivenza del sito e chiesto all'azienda di valutarlo. Si è evidenziato infine come la questione dello stabilimento di Battipaglia debba assumere rilevanza nazionale, essendo una delle poche aziende del Sud a portare avanti progetti significativi per l'intero settore delle La perdita delle competenze del sito rappresenterebbe pertanto una perdita per l'intero settore produttivo in Italia. Il Ministero dello sviluppo economico continuerà a lavorare assieme al Ministero degli affari esteri al fine di sensibilizzare i vertici dell'Alcatel-Lucent per

di consentire alle istituzioni di avere il tempo di percorrere le suddette strade. Un nuovo incontro per fare il punto su eventuali percorsi alternativi potrebbe essere quindi riprogrammato entro le prossime settimane.

qui stiamo parlando di una vicenda molto delicata e difficile, come la risposta del Governo ha già evidenziato e si desumeva anche dalla mia interrogazione. C'è una sofferenza notevole in un territorio già fortemente penalizzato per una serie di accadimenti che si sono verificati negli ultimi anni in tema di deindustrializzazione e dismissione dei livelli occupazionali, in un'area più complessiva, quella del salernitano, del battipagliese, della Piana del Sele e del Mezzogiorno, fortemente critica da questo punto di vista. parliamo di circa 200 lavoratori a tempo indeterminato, di altrettanti a tempo determinato e interinali per le attività di ricerca, sviluppo e produzione industriale nel settore delle trasmissioni ottiche,

il fatto che il Governo abbia prontamente posto in essere la convocazione di un tavolo interministeriale, chiamando a responsabilità anche livelli di Governo locale (la Regione, innanzitutto, e la Provincia, che aveva espresso - come spero confermerà - la propria disponibilità in questo senso). Il problema che

malgrado la crisi economica che attraversa l'intero Paese e tanta parte d'Europa e del mondo. Alcatel-Lucent vanta un portafoglio di prodotti di prim'ordine ed esprime una notevole capacità competitiva. La mia

è quanto chiedo al Governo, rendendomi interprete di questa forte e purtroppo fondata preoccupazione diffusa sul territorio tra le lavoratrici ed i lavoratori a qualunque titolo impegnati nella Alcatel. Alcatel. Bisognerà che il Governo spinga ancora, prima per il mantenimento e poi per il rilancio del sito produttivo di Battipaglia di Alcatel-Lucent, che tra l'altro ha realizzato un connubio eccellente anche con il mondo della ricerca e dell'innovazione, mettendo in atto una serie di collaborazioni anche con le università, in primo luogo con l'ateneo salernitano. Sarebbe veramente un peccato per il Mezzogiorno e sarebbe davvero deleterio per un'area già così tristemente afflitta dal

la società Po Valley e l'inizio dei lavori di perforazione nel parco di Montevecchia Valle del Curone. La Po Valley è una società italiana che fa capo ad una *holding* australiana; l'azienda opera nel settore dell'esplorazione e produzione di idrocarburi, prevalentemente nel Nord Italia che è, com'è noto, una delle aree più ricche di giacimenti di idrocarburi in Europa. Nel 2008 tale società ha presentato istanza per l'ottenimento di un permesso di ricerca di idrocarburi nella provincia di Lecco.

Allo stato attuale, in relazione al progetto Bernaga, non risulta siano state rilasciate autorizzazioni a procedere né dalle amministrazioni locali, né sicuramente dal Ministero dello sviluppo economico, pertanto nessun intervento è stato attuato o è in procinto di essere attuato sul territorio in questione. Quanto al progetto Ossola, si fa presente che lo scorso anno è stata avviata dal Ministero dello sviluppo economico l'istruttoria relativa ad una domanda di permesso avanzata dalla società Po Valley relativa allo stesso che interessava circa 300 in parte ricadenti nella provincia di Lecco. A seguito dell'avviso contrario all'iniziativa, espresso nelle conferenze dei servizi iniziali da molti dei Comuni interessati, l'istruttoria è stata subito sospesa. società, insieme con la società Edison, nel frattempo, ha riproposto la ricerca, su un'area molto ridotta (circa 30 chilometri quadrati), tutta in provincia di Lecco, ora denominata Bernaga. Conseguentemente, l'ufficio istruttore del Ministero dello sviluppo economico, tenuto conto delle opinioni già espresse dagli enti locali, con nota in data 5 maggio 2009, ha invitato i richiedenti a rivolgersi preventivamente agli enti locali per verificare la compatibilità ambientale dell'iniziativa, mantenendo sospesa l'istruttoria. In caso di mancato consenso locale, anche la nuova richiesta sarà archiviata. Si fa, comunque, presente che il processo di eventuale approvazione dell'istanza inoltrata dalla Po Valley richiede, per legge, dai 12 ai 18 mesi per l'effettuazione di analisi tecnico-ambientali e di consultazione con le comunità locali. Nel ribadire che, al momento, non vi è alcuna ipotesi di assegnazione di permessi ed autorizzazioni a perforare, si precisa che la stessa società Po Valley ha reso noto di essere intenzionata a portare avanti l'istanza di richiesta di permesso di ricerca in totale trasparenza e aprendo un dialogo onesto e cooperativo con le comunità locali coinvolte. In ogni caso, il Ministero dello sviluppo economico assicura che, qualora fosse conferito un permesso di ricerca, non sarebbero consentite perforazioni in aree del parco della Valle del Curone, né altre attività esplorative, salvo quelle espressamente autorizzate dall'ente parco stesso.

non poche preoccupazioni a livello territoriale, provinciale e tra i Comuni interessati di Rovagnate e di Olgiate, che ricadono all'interno

pareri e giudizi in merito a determinate operazioni, che vanno ad intaccare un ambito da anni tutelato dal punto di vista paesaggistico

dell'interesse generale e delle normative nazionali che giustamente devono tutelare la ricerca di fonti energetiche (in questo caso, di idrocarburi), le realtà locali, che sono le prime sentinelle dei nostri territori.

a parole; lo si deve attuare e questo Governo deve esserne rispettoso nei fatti. C'è una ambiguità che vorrei fosse espulsa dalla sua risposta, zona di così grande pregio anche operazioni di studio e di ricerca o, come lei le ha chiamate, di esplorazione, che comportino prove di trivellazione e scavi.

un'area tutelata da numerosi vincoli paesaggistici e ambientali ed esclusa da qualsiasi attività di tipo produttivo. Già l'ENI dieci anni fa aveva scartato qualsiasi ipotesi di trivellazione perché affermava che gran parte dell'area di studio è soggetta a vincoli idrogeologici, compreso il sito di perforazione. Inoltre, il Ministero dell'ambiente nel giugno del 2001 aveva dato parere negativo in considerazione «delle molteplici problematiche ambientali che la realizzazione del pozzo di ricerca comporterebbe, collocandosi all'interno di un area confinante con il pregiato Parco regionale di Montevecchia e della Valle del Curone» e «del disagio che la realizzazione del progetto comporterebbe per la comunità e per l'ambiente in termini di inquinamento acustico e atmosferico, nonché per le interferenze negative sulla flora e sulla fauna». Ho colto positivamente, signor Sottosegretario, l'intenzione da parte del soggetto proponente l'attività di ripristinare il dialogo con gli enti locali. Forse andava iniziato prima, non c'era bisogno di ripristinarlo solo dopo le risposte perentorie degli enti locali. Mi auguro anche che

Infatti, - riprendo le sue parole - un vero federalismo non può non partire dalle autorizzazioni e dalle risposte delle comunità locali che hanno la prima parola al riguardo.